ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del parere della Giunta per il Regolamento espresso nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Siciliana, a seguito delle dimissioni del senatore Salvatore Cuffaro, ha riscontrato, nella seduta di Salvatore Cuffaro, ha riscontrato, nella seduta di ieri, che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva il predetto senatore è Maria Giuseppa Castiglione. Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e proclamo senatore la signora Maria Giuseppa Castiglione, alla quale auguro buon lavoro. Avverto Avverto che da oggi decorre, nei confronti della nuova proclamata, il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami.

recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», introduce il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato ai sensi del quale lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione «è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro»; nel corso dell'esame al Senato in prima lettura, era stato approvato un emendamento della Lega Nord soppressivo del comma 5 dell'articolo 35 del testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo al divieto per le strutture sanitarie di denunciare all'autorità lo straniero non in regola con le norme sul soggiorno, salvo i casi in cui fosse obbligatorio il referto; il il suddetto articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - fortunatamente reintrodotto, grazie al lavoro dell'opposizione, nel corso dell'esame del disegno di legge alla Camera dei deputati - nel rispetto del principio costituzionale di tutela

Le nostre Madri e Padri costituenti certamente avranno riflettuto sull'utilizzo del sostantivo «individui» invece della parola «cittadini», che è utilizzata in molte altre parti della nostra Carta costituzionale.

il diritto alla salute, o meglio, il diritto alle cure, è un diritto per tutte le persone presenti sul territorio nazionale: non solo dei cittadini, ma anche degli immigrati, seppure irregolari. La soluzione normativa scelta, in vigore dal 1999 al 2009 (quindi per circa anni), oltre ad assicurare il rispetto di un diritto fondamentale, ha consentito la possibilità di curare quegli immigrati che, a causa delle loro condizioni di salute, hanno deciso di manifestarsi e di lasciare emergere la propria condizione di irregolarità, con il conseguente vantaggio di impedire un loro peggioramento, dannoso per l'individuo

se non volevano andare in questa direzione per generosità, lo avrebbero dovuto fare per egoismo, perché una persona che, ad esempio, è infetta da un microrganismo, come quello che provoca la tubercolosi, se non si avvia a un centro di cura certamente rimarrà

in capo al personale sanitario resta comunque una facoltà di denuncia. La risposta va trovata con specifico riferimento all'articolo 365 del codice penale; questa disposizione sanziona la «Omissione di referto». Questa norma si pone in un rapporto di specialità con i precedenti articoli 361 («Omessa denuncia da parte di pubblico ufficiale») e 362 («Omessa denuncia da parte di incaricato di pubblico servizio»), perché individua esattamente il soggetto attivo che è l'operatore sanitario;

che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516»; l'articolo 362 del codice penale («Omessa «L'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103»; tornando al rapporto di specialità risulta quindi evidente come, facendo l'articolo 365 del codice penale riferimento specifico al personale sanitario, si applichi questa disposizione rispetto a quella più generica prevista dall'articolo 361 del codice penale relativa alla figura più ampia ed indistinta dei pubblici ufficiali; inoltre, poiché l'articolo 365 del codice penale fa espresso riferimento al delitto come fattispecie che il personale sanitario ha l'obbligo di denunciare qualora ne venga a conoscenza, appare evidente come, essendo il reato di immigrazione clandestina classificato come una contravvenzione (per la quale è prevista un ammenda da 5.000 a 10.000 euro) e non come un delitto, l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, previsto per le strutture sanitarie dall'articolo 365 del codice penale, viene meno, essendo appunto previsto solo per i delitti; escluso infatti che, al di fuori dei casi di cui all'articolo 365 del codice penale, non ci sia un «dovere» di denuncia, non c'è neanche la facoltà. Ed è, infatti, proprio la facoltà di denuncia che il comma 5 dell'articolo 35 del testo unico sull'immigrazione da quanto esposto si comprende facilmente come non ci sia un'interpretazione univoca delle norme in esame, al punto che alcuni giuristi ribadiscono che l'introduzione del reato di immigrazione clandestina contenga in sé comunque l'obbligo per il personale sanitario, in quanto pubblico ufficiale, di denunciare l'immigrato irregolare, non tenendo conto quindi del rapporto

al fine di non creare confusione al personale sanitario, medico e non medico, tenuto a svolgere il proprio lavoro in tranquillità, garantendo il diritto alla salute di tutti coloro che hanno bisogno di essere curati, a prescindere dal loro status di «regolarità», si chiede di sapere: quali siano stati, in questi mesi, gli effetti e le conseguenze dell'introduzione nell'ordinamento del reato di immigrazione clandestina relativamente al ruolo ed agli obblighi per il personale sanitario, medico e non medico, nell'esercizio e a causa delle sue funzioni ed alle modalità di accesso dei cittadini extracomunitari ai centri di pronto soccorso; se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare ogni iniziativa utile a chiarire l'effettiva portata applicativa della disciplina relativa al reato di immigrazione clandestina, al fine di evitare che il personale sanitario, medico e non medico, svolga il proprio delicato e fondamentale lavoro con il dubbio, nel momento in cui il paziente sia un cittadino extracomunitario, di commettere un reato e di poter essere oggetto di sanzioni; quali iniziative urgenti intenda altresì adottare per continuare ad assicurare a chiunque, senza dubbio alcuno, il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute quale ambito inviolabile della dignità umana, come indicato all'articolo 32 della Costituzione e più volte ribadito dalla Corte costituzionale. **Saluto ad una rappresentanza

i senatori che hanno sottoscritto l'interpellanza o l'interrogazione, i senatori che sono interessati e il rappresentante del Governo che risponde.

pur introducendo il reato contravvenzionale di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato al suo articolo 1, comma 16, non ha in effetti apportato alcuna modifica all'impianto normativo del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione), in materia di tutela sanitaria dei cittadini extracomunitari non in regola con le norme inerenti al soggiorno: l'articolo 35 del decreto legislativo n. 286 del 1998 è rimasto invariato. Pertanto, ai sensi del comma 5 della norma in argomento, a favore dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno sono previsti tre distinti settori di intervento, ed esattamente: cure ambulatoriali urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio; cure ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio; interventi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. In particolare, sono garantiti: la tutela sociale della gravidanza e della maternità; la tutela della salute del minore; le vaccinazioni previste dalle vigenti disposizioni; gli interventi di profilassi internazionale; la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive. Si segnala inoltre che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 35 del suddetto Testo unico, l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non deve comportare alcun tipo di segnalazione da parte del personale sanitario, medico e non, alle autorità di pubblica sicurezza, salvi i casi per cui sia obbligatorio il referto, così come si verifica nelle stesse condizioni per il cittadino italiano. A tal riguardo, la circolare 27 novembre 2009, n. 12, diramata dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha inteso espressamente precisare che il comma 5 dell'articolo 35 prevede, per tutto il personale che opera presso le strutture sanitarie, il divieto di segnalazione all'autorità dell'accesso alle prestazioni sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno, salvi i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano. Con la medesima circolare è stato altresì fatto presente che l'obbligo di referto, disciplinato all'articolo 365 del codice penale, sussiste in presenza di delitti per i quali si deve procedere d'ufficio e che quindi, nel caso di reato d'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, tale obbligo non sussiste, stante la natura contravvenzionale e non di delitto Si evidenzia altresì che il comma 2 dell'articolo 365 del codice penale esclude espressamente l'obbligo di referto nell'esercizio di una professione sanitaria nel caso in cui il referto stesso possa esporre l'assistito a procedimento penale.

di soggiorno nel nostro Paese che si avviano per problemi di salute alle nostre strutture del Servizio sanitario nazionale,

bambini, donne e uomini dalle cure che il Servizio sanitario nazionale può offrire loro, mettendo a rischio la loro vita di fatto, una ferita alle norme del nostro ordinamento, in particolare all'articolo 32 della nostra Costituzione. Tali

per paura non si reca ad un pronto soccorso e sale invece sulla metropolitana di Milano evidentemente crea un pericolo per tutta la popolazione.

Con la scelta operata, la stessa persona viene a cumulare tale incarico con quello di presidente dell'Istituto superiore di sanità. La scelta di collocare la stessa persona al vertice di due importanti organismi, probabilmente i più importanti, preposti alla tutela della salute appare non motivata. La somma di incarichi e responsabilità quali quelli sopra indicati può esporre i citati organismi a un *deficit* di funzionalità, efficienza, produttività, ad un conflitto di interesse, come nella recente vicenda che abbiamo tutti avuto modo di leggere sui quotidiani negli ultimi dieci giorni, riguardante un dubbio sulla sicurezza o non sicurezza degli emoderivati che vengono utilizzati nel nostro Paese. Ad un certo momento del dibattito e del confronto istituzionale, l'Istituto superiore di sanità che, appunto, è presieduto dal professore Garaci ha dato un suo importante e autorevole parere sulla sicurezza dell'utilizzo di questi emoderivati nel Paese. Il Ministro giustamente, come è previsto dell'ordinamento, si è rivolto al Consiglio superiore di sanità per chiedere un'opinione su quanto aveva espresso

penso che sia un problema piuttosto importante, dal momento che riguarda la salute pubblica di tutte le persone che si rivolgono al Servizio sanitario nazionale e, in quel caso, devono con sicurezza essere sottoposti all'infusione di un prodotto emotrasfusionale. si chiede di sapere se e come siano state valutate altre possibili candidature alle due cariche e per quali vie si sia appurata la maggiore appropriatezza e corrispondenza del professor Garaci all'incarico ricevuto rispetto ad altre ipotesi nominative individuabili nella platea di eccellenti scienziati che l'Italia vanta per ruoli di alto livello e responsabilità.

Recentemente l'Istituto per la competitività, che annualmente stila una classifica, ha valutato quali siano, sulla base del cosiddetto *citation index*, i nostri 20 scienziati migliori, quelli che vengono chiamati nelle riviste internazionali i 20 *top scientists*. I nostri 20 *top scientists*

in Italia, o tra gli italiani all'estero, nessun altro in grado di ricoprire almeno una delle due cariche oggi occupate dal professor Garaci medesimo e se la comunità scientifica non debba leggere dall'accaduto il messaggio di una pratica politica che effettivamente odora di chiara lottizzazione e che esalta il merito di una sola persona, dimenticando volutamente altri scienziati, del cui valore il Ministero della salute avrebbe potuto giovarsi per politiche di tutela della salute in grado di soddisfare un diritto costituzionalmente garantito.

il decreto ministeriale n. 342 del 6 agosto 2003, e successive modifiche e integrazioni, disciplina la composizione del Consiglio superiore di sanità, stabilendo, all'articolo 1, comma 3, che il medesimo è costituito da membri non di diritto, nominati dal Ministro della salute,

preposti ai dipartimenti ed alle direzioni generali del Ministero della salute, dal presidente dell'Istituto superiore di sanità, dal presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, dal direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari Sono, altresì, componenti di diritto del Consiglio superiore di sanità il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, il presidente del Comitato scientifico permanente del Centro per il controllo delle malattie il presidente della Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri (FNOMCeO), il presidente della Federazione ordini farmacisti italiani (FOFI), il presidente della Federazione nazionale collegi infermieri (IPASVI) e il presidente della Federazione nazionale collegi ostetriche Occorre sottolineare che i componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità sono nominati in ragione della loro particolare qualificazione nelle materie attinenti alle competenze istituzionali del Consiglio stesso. Si tratta, invero, di valutazioni effettuate su base curriculare, che nulla hanno a che vedere con i particolari e personali orientamenti politici propri di ciascun individuo. D'altra parte, appare chiaro che l'equilibrata sintesi e rappresentanza dei diversi orientamenti della società civile e scientifica non si misurano dal grado di affezione o disaffezione ad un determinato schieramento politico, ma dalla idoneità dei singoli membri prescelti a rispecchiare e rappresentare le differenti competenze presenti nell'attuale comunità scientifica, con precipuo riferimento ai problemi di salute pubblica più rilevanti, con cui il Consiglio superiore di sanità è chiamato a confrontarsi. Venendo alla nomina del professor Enrico Garaci quale presidente del Consiglio superiore di sanità, occorre sviluppare alcune considerazioni. In primo luogo, va evidenziato che la carica di presidente del Consiglio superiore di sanità è una carica elettiva, conferita, pertanto, dall'organo stesso, mediante ordinaria votazione. Nel caso specifico, il professor Garaci è stato eletto, su proposta del professor Garattini, per acclamazione dal *plenum* dell'organo consultivo, con esplicito riconoscimento delle sue altissime qualità scientifiche ed esperienze in ambito universitario, clinico e di ricerca. Nel corso della riunione di insediamento del Consiglio superiore di sanità è stata proprio messa in luce l'idoneità del profilo del professor Garaci a coniugare conoscenza clinica, esperienza di ricerca scientifica, esperienza in epidemiologia, nonché l'altissima capacità istituzionale mostrata, in particolare, nel rivestire la carica di presidente del Consiglio superiore di sanità nel semestre precedente. Va riconosciuto, infatti, che egli è stato per più di dieci anni il rettore fondatore dell'università di Roma Tor Vergata, nonché presidente del Consiglio nazionale delle ricerche ed ha al suo attivo un'intensa attività di ricerca, documentata da pubblicazioni di elevato impatto scientifico. D'altra parte, il fatto che il professor Garaci sia presidente dell'Istituto superiore di sanità non è ostativo alla sua elezione a presidente del Consiglio superiore di sanità: non lo è dal punto di vista giuridico, né può esserlo sotto un profilo di mera opportunità, dal momento che può sviluppare una più consapevole sinergia tra le due istituzioni. Inoltre, anche in considerazione della fase di transizione e trasformazione che sta attraversando il Consiglio superiore di sanità, deve essere a nostro avviso valutata con favore la scelta operata dall'assemblea di attribuire la presidenza ad una personalità di rilievo

è parlato di "equilibrata sintesi". Certamente non saprei immaginare una sintesi migliore di quella di mettere la stessa persona a capo delle due più importanti istituzioni che controllano la sanità pubblica nel nostro Paese. Sono sicuro

dell'etica pubblica nelle nostre azioni. È evidente, infatti, che in questo caso non si tratta di fare un'analisi del *curriculum vitae* del professor Garaci, ma si tratta di stabilire se ognuno di noi, nell'esercizio delle proprie funzioni, ritiene che dal punto di vista etico sia corretto

appartenga alla propria etica personale la decisione, ad esempio, di dimettersi da una delle due cariche. Penso anche che il nostro Paese abbia davvero bisogno, un disperato bisogno, di dare

quel che ha detto il Sottosegretario, dal punto di vista legale, è corretto e legittimo, ma dal punto di vista pratico dà ancora una volta l'immagine di un Paese che si arrocca dietro le regole e le norme e che non è capace di fare quel passo

sul carattere esclusivo del rapporto di lavoro riguardante i direttori scientifici dell'IRCCS** il 16 ottobre 2003 è stato emanato il decreto legislativo n. 288 riguardante il «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. l'articolo 1 del citato decreto legislativo stabilisce che «Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti (...) che, secondo standards di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità»; attualmente in Italia sono 43 Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) che beneficiano di finanziamenti pubblici stanziati sia per la ricerca scientifica corrente, sia per la ricerca finalizzata, ma la cui erogazione avviene di fatto su basi discrezionali in assenza di un sistema rigoroso di valutazione scientifica dei risultati;

Le funzioni di direttore sanitario e di direttore amministrativo cessano al compimento del sessantacinquesimo anno di età»; nel dicembre 2006, nel corso della discussione parlamentare e dell'esame degli emendamenti relativi alla legge finanziaria per il 2007, l'Aula del Senato approvò un emendamento a firma del primo firmatario della presente interpellanza e del senatore Giovanni Legnini, il cui testo recitava: «La natura esclusiva degli incarichi del direttore generale, del direttore scientifico, del direttore amministrativo e del direttore sanitario degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, comporta l'incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l'esercizio di qualsiasi attività professionale»; il ricordato emendamento divenne il comma 820 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007; considerato, inoltre, che si registrano casi di violazione delle citate norme di legge sulla esclusività del rapporto di lavoro in caso di conferimento di incarichi direttivi e scientifici presso gli IRCCS, con l'interpellanza si vuole sapere se risultino al Ministro, attualmente in carica, presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, direttori scientifici che cumulino detto incarico con altri rapporti di lavoro variamente denominati con realtà, istituzioni e soggetti esterni agli IRCCS medesimi; se risultino incarichi di direttore scientifico presso presidi ospedalieri classificati come IRCCS cumulati con incarichi conferiti da università; se non si ritenga che l'importanza, la delicatezza e le attese che suscita tra i ricercatori, gli scienziati, nella pubblica opinione un'attività come la ricerca biomedica richieda un'attenzione più vigile verso una scrupolosa osservanza delle norme sull'esclusività richiesta per ricoprire fondamentali incarichi in strutture che devono produrre ricerca, risultati, eccellenza scientifica, competitivi ai più alti livelli e internazionalmente apprezzati; se non sia opportuno e doveroso scongiurare e deprimere ogni propensione a produrre «sanatorie», pratica annosa che, a nostro avviso, ha prodotto solo guasti. Mi chiedo, e le chiedo, se, in questa stessa ottica, non sia da ribadire esplicitamente che non sono ammesse autorizzazioni in deroga a quanto il Parlamento ha stabilito, perché ciò compromette la produttività scientifica degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; se l'eventualità di una «sanatoria» attraverso una legge che renda possibile la non esclusività nel rapporto di lavoro dei direttori scientifici degli IRCCS non sia in contraddizione aperta con l'esigenza di dotare codeste

in merito alla questione del cumulo di incarichi dei direttori scientifici in carica presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), riguardo ad ulteriori rapporti di lavoro con altre istituzioni o con università, si precisa che il vigente quadro normativo ed, in particolare, l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dispone che nelle fondazioni e negli istituti non trasformati in fondazioni l'incarico di direttore scientifico è di natura autonoma ed esclusiva, con una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. La citata disposizione di legge ha affermato, quindi, la natura esclusiva dell'incarico di direttore scientifico presso gli IRCCS pubblici e, conseguentemente, l'incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato e con l'esercizio di qualsiasi attività professionale. Sulla esclusività dell'incarico di direttore scientifico presso gli IRCCS pubblici si è pronunciato anche il Consiglio di Stato - sezione prima - che, con parere reso nella adunanza del 12 ottobre 2005, ha evidenziato che «(...) l'esclusività del rapporto di lavoro del direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico figura apicale al pari del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario, tutte accomunate dalla identica disciplina di *status* prevista dall'articolo 11, del decreto legislativo n. 288 del 2003 - è prevista, allo stato, in modo così chiaro e tassativo, da non poter tollerare eccezioni o temperamenti di sorta, possibili solo attraverso una modifica della normativa vigente». Il Ministero della salute-Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica, pertanto, con lettera circolare del 14 settembre 2006 inviata agli IRCCS pubblici, ha invitato i responsabili della gestione degli stessi ad assicurare l'osservanza dei princìpi contenuti nel suddetto parere, ricevendone il positivo riscontro. L'osservanza della esclusività dell'incarico di direttore scientifico presso gli IRCCS è rimessa ai direttori generali degli stessi, con i quali però viene stipulato il contratto per l'espletamento dell'incarico in questione.

Agli atti della citata direzione generale, che esercita una funzione di vigilanza sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, non risulta, attualmente, che vi siano direttori scientifici presso IRCCS pubblici che svolgano altre attività lavorative: qualora il Ministero della salute venisse in possesso di elementi che potessero far emergere situazioni di incompatibilità, si assicura il pronto intervento sugli organi competenti per la cessazione di tali situazioni. Per quanto riguarda il riferimento all'eventualità di una "sanatoria" normativa che renda possibile la non esclusività nel rapporto di lavoro dei direttori scientifici degli IRCCS, è opportuno precisare che il principio dell'esclusività di detto rapporto non verrebbe meno nel caso in cui il direttore scientifico collaborasse con altre istituzioni medico-scientifiche o enti finanziatori della ricerca, senza pregiudicare la propria attività istituzionale. È necessario, pertanto, che tali collaborazioni non assumano la natura di rapporto di lavoro e prevedano esclusivamente un gettone di presenza per quanto riguarda le spese sostenute e l'utilizzo del tempo extralavorativo impiegato, come avviene, peraltro, per analoghe figure professionali dipendenti presso pubbliche amministrazioni. A titolo di esempio, le revisioni dei progetti inviati da amministrazioni pubbliche o da enti finanziatori o da centri internazionali di ricerca, non prefigurando alcun tipo di rapporto lavorativo, ma la semplice espressione di un'alta competenza nella materia scientifica, sono da considerarsi del tutto funzionali all'attività di direzione scientifica di un ente, attività che si identifica anche nel reperire fondi per la ricerca in ambito nazionale ed internazionale. È da rilevare, inoltre, che tali collaborazioni consentirebbero all'IRCCS sia di avvalersi dell'accresciuta professionalità del direttore scientifico sia di poter interagire, al fine di sviluppare ed ampliare in ambito nazionale ed internazionale i temi della ricerca, con il mondo scientifico del quale, proprio in tal modo, l'IRCCS ed il direttore scientifico risulterebbero essere parte integrante. [MARINO

tra le 43 figure che ricoprono il ruolo di direttore scientifico nel nostro Paese ve ne sono alcune che hanno altri incarichi, altri contratti lavorativi: se, ad esempio, sono presidi di facoltà, rettori o professori ordinari, oppure hanno altri incarichi incarichi lavorativi con contratti con altre istituzioni. Questo, lo dico con molta franchezza. Credo che vi siano Paesi che non si offenderebbero ad essere definiti capitalisti, come gli Stati Uniti d'America, dove chi assume il ruolo di direttore scientifico di un istituto di ricerca fa soltanto quel lavoro perché accetta con passione di dedicarsi interamente, per quella fase della sua vita, alla ricerca scientifica e alla direzione di un *team* di ricerca: lavoro straordinariamente appassionante, ma anche veramente molto impegnativo. Penso che nel nostro Paese vi siano invece dei direttori scientifici di alcuni dei nostri IRCCS che svolgono anche altri tipi di attività e professione, in questo modo distraendo il loro tempo da quello che è l'obiettivo principale, cioè la missione scientifica e l'eccellenza clinica. Dal momento che non ho ricevuto risposta se questo sia vero o no, e quindi rimango con questo dubbio (la Sottosegretario ha detto che se loro ne verranno a conoscenza sicuramente interverranno, però loro sono il Governo, e insomma dispongono dello strumento principale di controllo sul Servizio sanitario nazionale), chiederò, come membro della Commissione

da ocratossina arrivato al porto di Bari, il Ministero della salute assicura che sono stati adottati tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire la sicurezza del consumatore. Infatti, è stato attivato il sistema di allerta rapido comunitario sul territorio nazionale e si è proceduto all'acquisizione della rete di commercializzazione del grano contaminato da parte delle Regioni interessate, coadiuvate dai reparti dei NAS dei carabinieri, con il supporto tecnico dell'Istituto superiore di sanità; sono state tempestivamente attivate le procedure di rintraccio nel territorio della partita di grano incriminata e dei prodotti trasformati. Sono stati, altresì, intensificati i controlli all'importazione su tutte le partite dì grano provenienti dal Canada, da parte dagli uffici periferici del Ministero della salute. Relativamente alle misure da adottare per impedire che prodotti importati e destinati ad altro uso vengano fraudolentemente utilizzati per usi alimentari, si segnala che i sistemi di controllo in frontiera prevedono una documentazione di di importazione ed un provvedimento di ammissione della merce nel quale è indicata anche la destinazione d'uso dichiarata sotto la responsabilità dell'importatore. Tale documentazione accompagna la partita sino a destinazione finale e quindi può essere, in qualsiasi momento, controllata dalle Regioni e dalle ASL competenti per territorio, nonché dai vari organi di controllo di polizia.

Per quanto riguarda l'attivazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, comma 356, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA), in virtù dei particolari compiti ad esso affidati, ha assunto la denominazione di Autorità nazionale per la sicurezza alimentare con sede istituzionale presso il Ministero della salute e con la previsione di una sede referente operante presso la città di Foggia. In seguito, con l'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31 la citata norma della legge finanziaria è stata sostituita per cui la predetta Autorità nazionale per la sicurezza alimentare è stata trasformata, a decorrere dal 15 gennaio 2008, in Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, con unica sede in Foggia, posta sotto la vigilanza del Ministero della salute. Tale norma prevedeva, altresì, l'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per definire l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia medesima; tale provvedimento non è stato adottato. L'ente in questione, ancorché mai costituito, è inevitabilmente rientrato tra gli enti soppressi, ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 agosto 2008, n. 133. In base a detta disposizione sono stati soppressi tutti gli enti pubblici non economici per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non sono stati emanati i regolamenti di riordino, ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 con conseguente comunicazione, nei successivi 90 giorni, da parte dei Ministri vigilanti Si ritiene necessario, tuttavia, chiarire

Infatti, il comma 2, dell'articolo 26 della legge n. 133 del 2008 stabilisce che le funzioni esercitate dagli enti soppressi ai sensi del comma 1 della stessa norma sono attribuite all'amministrazione vigilante o a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. Detta amministrazione, inoltre, succede a titolo universale all'ente soppresso e ne acquisisce le eventuali risorse finanziarie, strumentali e di personale. Pertanto, le competenze dell'Agenzia restano attribuite al Ministero della salute, in cui era stata incardinata dalla legge n. 244 del 2005, il quale costantemente assicura, in attuazione degli obblighi comunitari che impegnano il nostro Paese, il coordinamento delle funzioni in materia di valutazione del rischio della catena alimentare. Per gli aspetti di competenza, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha inteso segnalare le attività espletate dal proprio organo di controllo, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, il quale ha il compito di prevenire e reprimere gli illeciti nei vari settori nel campo agroalimentare, compresi i mezzi tecnici di produzione agricola. I controlli svolti dall'Ispettorato consistono in ispezioni (condotte attraverso verifiche ed accertamenti, fisici e documentali) sulla conformità dei processi produttivi, sulla regolare tenuta della documentazione prevista dalla legge, sulla sussistenza ed idoneità dei sistemi di tracciabilità, sulla correttezza e veridicità delle informazioni riportate nell'etichetta L'Ispettorato, inoltre, provvede a svolgere controlli straordinari a sostegno delle produzioni agricole colpite da crisi di mercato; attuare controlli nelle filiere agroalimentari ove si siano manifestati o siano in atto andamenti anomali dei prezzi rilevati dall'osservatorio ministeriale; svolgere controlli diretti a contrastare l'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari; svolgere attività di coordinamento del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo delle capitanerie di porto, per l'attuazione delle azioni di controllo volte a tutelare la qualità delle produzioni agroalimentari e a contrastare le frodi in campo agroalimentare. Da diversi anni l'Ispettorato favorisce strategie rivolte ad incentivare forme di concorso con gli altri organi di controllo; sostiene la collaborazione con le Regioni e Province autonome; promuove la consultazione delle associazioni dei produttori e delle principali rappresentanze dei consumatori; dà impulso alla creazione di banche dati condivise tra le varie istituzioni incaricate del controllo, utili per potenziare gli scambi informativi e meglio indirizzarne l'attività di controllo. Per assicurare il coordinamento tra le diverse strutture coinvolte nei controlli in campo alimentare è operativo, presso l'Ispettorato, il comitato tecnico per il coordinamento delle attività di controllo nel settore agroalimentare. agroalimentare. Presieduto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il comitato riunisce i rappresentanti del Comando carabinieri salute (NAS), dei nuclei di polizia tributaria della Guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato, della Polizia di Stato, Comando carabinieri politiche agricole, del comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). In esito alle attività di controllo effettuate nel 2009 nel settore dei cereali sfarinati, pane e paste alimentari, sono stati riscontrati 74 prodotti irregolari, a fronte dei 3.325 prodotti sottoposti a controllo. Sono stati altresì analizzati 296 campioni, di cui 12 sono risultati irregolari. Per quanto riguarda le misure repressive irrogate, nel 2009 sono stati effettuati due sequestri, comunicate all'autorità giudiziaria tre ipotesi di reato e riscontrate 85 violazioni di natura amministrativa. I principali illeciti accertati, in particolare sugli sfarinati e sulle paste alimentari, riguardano l'irregolare tenuta dei registri di consegna e scarico relativi alle paste secche destinate all'esportazione; la commercializzazione di paste con parametri analitici difformi dai valori di legge (ceneri o umidità superiori); la commercializzazione, detenzione o impiego di pane, pasta e sfarinati aventi requisiti non conformi alle disposizioni di legge. L'attività di controllo viene diretta, oltre che sulla corretta commercializzazione dei prodotti agroalimentari nazionali (al fine di contrastare ogni forma di sleale concorrenza e consolidare la rinomanza dì tali produzioni, sia sul mercato interno sia in ambito comunitario e internazionale), anche su taluni prodotti provenienti da Paesi europei ed extraeuropei. Tale attività permetterà di contrastare più efficacemente la commercializzazione di prodotti esteri fraudolentemente etichettati di origine italiana, in modo da evitare situazioni di concorrenza sleale nei confronti degli operatori italiani e, contemporaneamente, di garantire la corretta informazione al consumatore finale circa l'origine dichiarata in etichetta.

Vorrei ricordare all'Assemblea che proprio la scorsa settimana abbiamo affrontato il tema della sicurezza alimentare, a seguito dell'allarme sulle carni alla diossina.

Vorrei ricordare alla Sottosegretario che, solo nei primi mesi del 2010, i NAS hanno sequestrato alimenti fuorilegge per circa 10 milioni di euro: il 40 per cento in più rispetto al primo semestre del 2009.

La Sottosegretario ha fatto riferimento ad un sistema di controlli, sia da parte del Ministero della salute sia da parte del Ministero dell'agricoltura. Voglio ricordare a noi tutti - e vengo al tema dell'Agenzia - che un conto è la gestione del rischio alimentare, un altro è la valutazione del rischio alimentare.

chi si occupa in Italia della sicurezza alimentare dei cittadini? Non mi riferisco alla repressione delle frodi, che è altra cosa: smettiamola di confondere i livelli.

questo. La Sottosegretario, poi, faceva riferimento ad una serie di norme che hanno portato alla soppressione dell'Agenzia. Ebbene, siccome l'emendamento non soppressivo porta la mia firma

al quale è stato possibile stabilire dove si era verificato il fenomeno, cosa che non è stato possibile fare con gli alimenti della Germania, di cui non sappiamo l'attuale diffusione in Italia e nel mondo. È vero che abbiamo il sistema di controlli migliore al mondo, però evidentemente c'è qualcosa che rende permeabile questo sistema,

Signor Presidente, la delocalizzazione delle emittenti, sia televisive che radiofoniche, site in San Silvestro di Pescara diviene un atto dovuto solo in presenza di un piano nazionale di assegnazione delle frequenze Tale piano è stato approvato il 15 giugno 2010 da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, mentre per le emittenti radiofoniche FM non si ha un piano nazionale. Ciò premesso, il sito ove delocalizzare gli impianti oggetto delle presenti interrogazioni era già stato individuato nel 2008 dalle ordinanze nn. 1 e 2 del Presidente della Regione Abruzzo nel sito di Pietra Corniale nel Comune di Bussi sul Tirino (Pescara), ovvero in altro sito, purché ritenuto idoneo sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni Un secondo sito citato dal piano è quello di Colonnella, situato in provincia di Teramo, avente un'area di servizio che comprende la costa da Martinsicuro a Francavilla, anch'esso non idoneo da solo, ma soltanto se utilizzato contemporaneamente a quello di Bussi sul Tirino. Gli impianti, quindi, dovrebbero essere distribuiti fra queste due località, ma, fermo restando la considerazione circa la drastica riduzione delle emittenti che potrebbero continuare a servire la città di Pescara ed il litorale, la nuova situazione di irradiazione imporrebbe ai cittadini, che oggi ricevono il segnale da San Silvestro, di installare nuovi impianti di ricezione, pena la perdita immediata del segnale all'atto dello spegnimento delle emittenti operanti da San Silvestro. In proposito occorre precisare che il Ministero dello sviluppo economico ha il dovere di garantire la continuità del servizio televisivo a tutela dei cittadini, soprattutto in considerazione del fatto che tra gli impianti da delocalizzare vi sono anche quelli del servizio pubblico, che è assoggettato a precisi obblighi di copertura. Proprio in tale ottica, il Ministero ha necessità di avere certezza che, anche con la delocalizzazione, sia possibile continuare a fornire ai cittadini - che ovviamente pagano un canone - la fruizione del servizio di radiodiffusione televisiva. Da ciò deriva la richiesta avanzata alla Regione Abruzzo di conoscere lo stato dei siti di Bussi sul Tirino e Colonnella, sia in termini di idoneità urbanistica, sanitaria e ambientale, sia di ricettività dal punto di vista della presenza delle infrastrutture. Si è ribadito, quindi, alla Regione Abruzzo l'invito a definire i piani territoriali sulla cui base vengono individuati i siti di trasmissione e a richiedere ai Comuni la disponibilità all'installazione degli impianti trasmittenti e lo stato di realizzazione delle infrastrutture necessarie all'attivazione dei trasmettitori è stato presentato uno studio di fattibilità per la delocalizzazione degli impianti radiotelevisivi presenti in San Silvestro su una piattaforma *offshore* prospiciente la costa abruzzese all'altezza di Pescara. Tale soluzione permetterebbe, secondo la Regione, di garantire la qualità del servizio di ripetizione del segnale nelle aree geografiche tuttora servite e nel contempo la risoluzione dei possibili rischi per la salute della popolazione residente. In data 13 gennaio si è tenuta una riunione della commissione consiliare permanente sanità del Comune di Pescara e in tale sede si sono fatti presenti gli inconvenienti che la soluzione di una piattaforma *offshore* presenta per i ripetitori TV e cioè: il disagio per l'utenza di dover variare l'orientamento delle antenne; l'eventualità, possibilmente da evitare, di una doppia variazione dell'orientamento, dovuta allo spostamento sulla piattaforma *offshore* degli impianti trasmittenti e l'ulteriore variazione nel passaggio al digitale, in quanto lo *switch-off* è previsto entro il corrente anno; la maggiore sensibilità, a causa del nuovo orientamento delle antenne TV, ai disturbi provenienti da trasmettitori allocati nei Paesi stranieri che si affacciano sull'Adriatico. Inoltre, gli operatori radiotelevisivi avranno, con tale allocazione, un aumento delle spese di manutenzione e gestione dei loro impianti. La commissione consiliare è orientata a dare parere favorevole al passaggio dei soli impianti radiofonici sulla piattaforma *offshore*, visto che per tali impianti non si hanno gli inconvenienti sopra elencati. In conclusione, si specifica che l'attività di vigilanza è stata garantita dagli ispettorati territoriali del Ministero e dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e che, in forza di quanto sopra esposto, il Ministero dello sviluppo economico è in attesa delle deliberazioni della Regione competente sul piano definitivo

Vi è un gravissimo pericolo immanente per la salute pubblica e un documentato rapporto di causalità tra l'esposizione ai campi elettromagnetici e l'insorgenza di gravi malattie, anche di tipo tumorale. Vi sono ormai molteplici casi che vengono denunciati e documentati. Per questa ragione, all'esito di numerose iniziative, ricorsi, procedimenti giurisdizionali, incontri, trattative, il Presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo, con l'ordinanza n. 1 del 24 giugno 2008, ebbe a disporre la delocalizzazione - come riferiva il sottosegretario Saglia - delle antenne degli impianti di radiodiffusione da questo ad altro sito. Da allora non è successo assolutamente nulla: anzi, ci risulta che l'*Authority* avrebbe deliberato recentemente, con l'atto n. 300 del 2010, una conferma di quella delocalizzazione, mentre la Regione Abruzzo - come ci ha detto il Sottosegretario - ritiene si debba realizzare una piattaforma *offshore* in modo tale da allontanare dall'abitato - certamente da San Silvestro, ma anche dal centro urbano di Pescara - quegli impianti. Ciò che rileviamo, in sostanza, è una sostanziale inerzia del Governo, una mancanza di impegno serio nell'affrontare e risolvere questo annoso problema e un rimpallo di responsabilità sempre più inaccettabile tra il Governo, la Regione e il Comune di Pescara. È certamente vero che bisogna tutelare il diritto dei cittadini utenti di vedersi raggiunti di vedersi raggiunti dalla comunicazione televisiva e radiofonica, ci mancherebbe altro: ma esistono soluzioni alternative, sono state proposte e dimostrate nel tempo, sono praticabili. Certo, comportano un costo; ma di fronte alla salute dei cittadini, così gravemente compromessa, e all'angoscia nella quale vivono centinaia e centinaia di famiglie che lì abitano stabilmente non non è possibile rinviare la soluzione di questo problema. Ecco la ragione per la quale torniamo a sollecitare il Governo, nella persona del sottosegretario Saglia, a promuovere con più determinazione, ferme le competenze sia del Governo che della Regione,

Per l'ennesima volta, tutta l'attività ispettiva del Parlamento viene costantemente mortificata da un'assenza del Governo nel dare risposte puntuali e specifiche. Su questo problema importante, importantissimo, come le ha ricordato il collega Legnini, noi dell'Italia dei Valori abbiamo infatti presentato una richiesta di chiarimento al Governo già nel giugno 2009, 2009, successivamente reiterata nel marzo 2010. Sono passati, onorevole Sottosegretario, quasi due anni, e le risposte che lei oggi ci ha dato sono assolutamente insufficienti e inadeguate ad affrontare un problema che cercherò di spiegare, in parole molto semplici, chiare e sintetiche, a chi ci sta ascoltando in questo momento. Un problema che può essere sintetizzato con la definizione che della collina di San Silvestro luogo di locazione e di accentramento di antenne elettromagnetiche - altri parlamentari prima di noi hanno dato: la collina della vergogna. Purtroppo, onorevole Sottosegretario, si tratta di una vergogna locale e nazionale, e le spiego perché. Locale, in quanto c'è un palleggiamento di responsabilità sulla pelle degli degli abitanti di quella zona che, con studi medici e scientifici, hanno dimostrato - a fronte delle preoccupazioni del Governo su chi deve avere un servizio pubblico RAI dopo il pagamento del canone - un aumento esponenziale delle malattie leucemiche, tumorali e di patologie da onde elettromagnetiche, al punto tale che alcuni di loro hanno dovuto intraprendere manifestazioni anche particolarmente forti ed eclatanti. Il palleggiamento di responsabilità è

del Consiglio europeo, votata all'unanimità l'anno scorso. Tale risoluzione invitava gli Stati membri a rivedere i livelli minimi e massimi di esposizione alle onde elettromagnetiche perché quelli attualmente previsti dagli Stati membri sono completamente superati dalle competenze e dalle indicazioni medico-scientifiche, in quanto il danno

Commissione europea e delle massime autorità scientifiche in materia, a stringere un rapporto di cooperazione interistituzionale con la Regione Abruzzo al

ricordando anzitutto che il presidente del Consiglio Berlusconi ha ormai una lunga esperienza nei rapporti internazionali e ha saputo ottenere rapporti

che hanno anche dato impulso a queste relazioni personali fondate su stima reciproca: l'azione dell'Italia per l'ingresso della Russia nel Consiglio NATO-Russia, il Vertice di Pratica di Mare del 2002, gli interventi dell'Italia per impegnarsi con altri importanti leader nel favorire una via d'uscita per la crisi Russia-Georgia, un'azione di sollecitazione verso la firma

l'introduzione di un principio fondamentale per l'Italia secondo il quale, nel considerare la situazione debitoria di uno Stato membro, oltre che del debito pubblico, tenere conto della situazione di sostenibilità complessiva del sistema Paese, quindi anche del risparmio e del debito privato. È evidente che tutto ciò si potrà proiettare anche in queste settimane complesse per una crisi del Mediterraneo, in cui l'Italia si sta adoperando. Vi sono contatti proprio in questi minuti tra i Capi di Governo di alcuni Paesi europei, tra cui l'Italia, per assumere una posizione forte e condivisa, da portare domani al Consiglio europeo, sulla difficile e estremamente preoccupante situazione in Egitto, al fine di auspicare una transizione rapida,

Certamente, abbiamo fatto molto a livello internazionale contro la criminalità organizzata. I sequestri di beni e di patrimoni per valori ingentissimi - oltre 16 miliardi di euro - hanno colpito fortemente i legami internazionali della criminalità mafiosa, con l'arresto di decine di pericolosissimi latitanti. È evidente che l'aver esteso il reato di associazione mafiosa alle organizzazioni criminali straniere ha comportato un grave danno - finalmente, voglio dire - a queste ramificazioni internazionali del crimine organizzato. L'Italia ha lavorato anche nella crescita dell'interscambio internazionale, più di quasi tutti gli altri Paesi europei: siamo secondi solo alla Germania, con un export che nello scorso anno è aumentato del 17 per cento. È un elemento importante, ed è altrettanto altrettanto evidente e chiaro che qualche denigrazione sistematica dell'Italia può avere un effetto negativo sul ruolo e sulle posizioni italiane, nel contesto di una competizione economica globale che non fa sconti, che è estremamente aggressiva e che profitta di ogni ipotesi e di ogni prospettiva, anche di attacco denigratorio all'immagine del Paese. In particolare, con riferimento al cuore della domanda posta dal senatore Zanda, vorrei assicurare che mai sono giunte, né direttamente, né indirettamente, tramite la rete diplomatica o per il tramite dei Servizi come ieri mi ha espressamente confermato per iscritto il direttore del Dipartimento informazioni per la sicurezza - delle ipotesi di valutazione raccolte all'estero circa una presunta ricattabilità del Presidente del Consiglio, né abbiamo avuto mai notizie di tentativi di forme di pressione in tal senso da parte di potenze straniere o, peggio, di organizzazioni criminali. Quindi, evidentemente l'Italia continuerà ad operare con l'impegno di sempre nei contesti internazionali, e raccogliamo frequentemente anche pubblici attestati dell'impegno, del ruolo del nostro Paese, in Europa e fuori dall'Europa.

della credibilità dell'onorevole Berlusconi. Debbo essere franco. Dagli atti trasmessi al Parlamento dall'autorità giudiziaria risulta che da anni il Presidente del Consiglio dei ministri è sottoposto ad un reticolo di pressioni, di piccoli e grandi ricatti da parte di persone della sua corte che lo frequentano e approfittano della sua ricchezza. Avrei voluto sentire dal Ministro parole chiare, che escludessero che un *leader* non solo sottoposto obiettivamente al ricatto di chi lo incontra, ma anche a vari procedimenti penali, imprudente nei costumi, in rapporto intimo con persone reclutate per lui da altri e introdotte nelle sue abitazioni senza alcun controllo di polizia, sia considerato dalla diplomazia internazionale persona esposta anche ai grandi ricatti di potenze straniere, Ho chiesto al Ministro informazioni sui giudizi informali

sull'affidabilità di un leader così platealmente soggetto a forme potenziali di ricatto. Avrei voluto sentire il Ministro degli esteri contraddire il ministro Bossi, che tempo fa ha sostenuto che nelle disavventure femminili di Berlusconi c'è la mano della mafia. Di ricatto di mafia ha parlato un Ministro della Repubblica, non io.

In un'intervista tempo fa lei ha detto che tutto si risolve in una sorta di curiosità dei Governi stranieri per il carattere esuberante del Premier. Lo ha detto lei. Oggi forse avrebbe potuto almeno ricordare i rapporti dell'ambasciata americana in Italia resi noti da WikiLeaks. Oppure avrebbe almeno potuto accennare ai giudizi morali della Santa Sede. Non è credibile che l'unica persona che non si accorge di quanto siano diffusi all'estero il fastidio e la preoccupazione per le conseguenze dei comportamenti di Berlusconi sia proprio il Ministro degli affari esteri italiano. Nella mia attività parlamentare ho sempre evitato, perché mi dà fastidio, di usare la parola "regime": ma oggi debbo usarla. Nei regimi non c'è solo la limitazione del potere legislativo, il controllo di tanta parte dell'informazione, l'influenza sulla grande finanza e l'occupazione di pezzi dello Stato: cose che conosciamo. Nei regimi c'è anche il culto del capo, la pretesa di una sua immunità totale e la copertura complice dei suoi vizi, anche di fronte all'evidenza dei fatti. Nei regimi, se il capo è accusato di favorire la prostituzione minorile, la sua corte dice che ha soltanto passato un'allegra serata. L'evanescente risposta del ministro Frattini conferma che le vicende di Berlusconi sono una sorta di sigillo del suo personale sistema di potere, nel quale, come in tutti i regimi, il pubblico e il privato, il politico e il personale si confondono, si intrecciano e si sorreggono a vicenda. Tutti, nell'*entourage* di Berlusconi, compresi i suoi colleghi di Governo e l'intero gruppo dirigente del suo partito, conoscevano da tempo i rischi dei suoi costumi privati e della disinvoltura con la quale apriva la sua casa a sconosciuti. Ma nessun membro del Governo, nemmeno oggi il ministro Frattini, ha mai sollevato la questione della possibile ricattabilità dell'onorevole Berlusconi. Questo silenzio è il segno più chiaro

Su richiesta dei Presidenti delle Commissioni 1a e 5a, i lavori in sede referente sul decreto-legge recante proroga di termini legislativi potranno proseguire fino a tutta la giornata di mercoledì 9 febbraio. Nel corso della prossima settimana si terranno due sedute. Mercoledì 9, alle ore 16, il Ministro dell'interno renderà un'informativa sulla regolarizzazione di lavoratori extracomunitari e sui flussi di ingresso. Successivamente potranno intervenire i rappresentanti dei Gruppi, per 5 minuti ciascuno. Giovedì 10 febbraio, alle ore 10, avrà inizio 1'esame del predetto decreto in materia di proroga termini, con lo svolgimento delle relazioni. Si passerà poi al voto di eventuali questioni incidentali e alla discussione generale. La seduta unica sarà sospesa dalle ore 14 alle ore 15. Il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti è stabilito per le ore 19 di giovedì 10 febbraio. La discussione del provvedimento riprenderà la settimana successiva, a partire dalle ore 12 di martedì 15 febbraio. Nel corso della stessa settimana saranno inoltre esaminati il decreto-legge recante proroga di missioni internazionali, già approvato dalla Camera dei deputati -per il quale si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi - e, se concluso dalla Commissione, il disegno di legge sulla parità di accesso